ha stabilito che il dibattito, comprensivo di relazioni, discussione generale ed esame degli emendamenti, avrà complessivamente la durata di tre ore. In relazione al numero di emendamenti e ordini del giorno presentati, i tempi sono stati così ripartiti:

Ai fini del buon andamento dei nostri lavori, si ricorda che le dichiarazioni di voto inizieranno in ogni caso alle ore 14, essendo prevista la trasmissione diretta televisiva. Ilrelatore, senatore Malan, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

le parti del provvedimento, nel testo approvato dal Senato, che sono state soppresse nel passaggio presso l'altro ramo del Parlamento. È stata soppressa la norma che prevedeva la sospensione della demolizione di

così come due norme riguardanti la riorganizzazione della CONSOB. È stata inoltre soppressa una norma riguardante le modalità di rilascio dei brevetti per il salvamento acquatico; è stata soppressa

una norma tesa a modificare la proroga del Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici,

è stata lievemente modificata una norma approvata in Commissione riguardante le valli da pesca della laguna di Venezia. riferimento infine alle disposizioni concernenti il sistema bancario originate dall'inserimento di un articolo nell'emendamento presentato dal Governo in Aula, sul quale è stato posta la fiducia, è stata aggiunta una norma riguardante l'interpretazione dell'articolo 2935 del codice civile relativo all'anatocismo con cui si specifica che, in ogni caso, non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

il Presidente del Consiglio appena due giorni fa aveva manifestato una critica al Parlamento, censurandolo per il fatto che le iniziative legislative

Siamo stati insomma rimproverati: la maggioranza, in modo particolare, è stata rimproverata di stravolgere le intenzioni del Governo. A distanza di 24 ore, il Governo avrebbe avuto la possibilità di trasformare l'ippopotamo in puledro di razza, ossia di ripulire il decreto‑legge, così come ideato dal Governo e stravolto dall'iniziativa parlamentare, appesantito enormemente. Il Governo, specie dopo il richiamo del Capo dello Stato contenuto nella lettera che lei, signor Presidente, ci ha letto in Aula, aveva questa possibilità enorme di dimostrare subito come si può tornare ai puledri di razza.

le materie non contenute nel testo originario e che continuano ad avere una qualche disciplina nel nuovo testo proposto dal Governo sono in numero di 103: rispetto al puledro licenziato dal Governo con il decreto originario, vi sono materie nuove, proposte con l'emendamento del Governo, in numero di 103. In questo modo, non penso che si sia data una risposta ai profili di costituzionalità sottolineati nella lettera del Presidente della Repubblica. Continuano a rimanere afflitte da vizio tutte quelle proroghe che vengono così disciplinate: per un primo periodo di proroga, si interviene con legge ordinaria, ma si ma si prevede che per un successivo periodo di proroga si possa intervenire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In una legge viene prorogata nei termini con due atti aventi natura diversa: uno, avente rango legislativo; l'altro, avente rango amministrativo. Questa è una profonda contraddizione. un'altra profonda contraddizione che si ricava dalle proposte che ci apprestiamo a votare.

viene anticipato al 31 marzo 2011, con possibilità di proroga al 31 dicembre 2011. Con questa proroga si conferisce al Presidente del Consiglio dei ministri la potestà di prorogare, ovvero di non prorogare, il divieto di acquisto di quotidiani per chi eserciti attività televisiva con più di una rete. In altri termini, il Presidente del Consiglio dei ministri valuterà fino a quando un'impresa, anche quella che fa capo a lui stesso, potrà o non potrà eventualmente acquisire quotidiani nazionali.

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con nota del 24 novembre 2010, avesse espressamente sollecitato l'opportunità di mantenere in vigore il divieto di cumulo previsto dalla legge

ed etici. Colleghi, ditemi se è etico che la proroga del pagamento delle sanzioni per le quote latte, ulteriormente ampliata, preveda una copertura di 5 milioni di euro

per l'assistenza ai malati terminali. Questa è la più grave offesa che potesse farsi al Paese, all'etica e alla morale!

di non procedere, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, all'esame di questo atto. dobbiamo confrontarci con la nota metafora del Presidente del Consiglio

Ora, è uscito dal Consiglio dei ministri un destriero marchiato «destriero» o c'era già scritto «ippopotamo»? Secondo me c'era già scritto ippopotamo, perché l'ispiratore del titolo di questo decreto, che poi condiziona le ammissibilità,

«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie». Con un titolo del genere, si nasce ippopotami, perché quasi tutto diventa ammissibile; quindi il Presidente del Consiglio, invece di prendersela con il Parlamento, se la prenda con il suo Governo, perché è lui che crea ippopotami, non il Parlamento. Il Parlamento ci può mettere del suo e peggiorare, ma c'era già scritto ippopotamo, non c'era scritto destriero Quando uno fa un decreto del genere, sa già che sarà un *soufflé* destinato a lievitare in maniera inconsulta; tanto più se lo fa dopo che, dall'inizio della legislatura, il Presidente della Repubblica ha richiamato più volte sulla rigidità dei criteri di ammissibilità degli emendamenti parlamentari sui decreti, in modo da evitare di andare ad incidere sul controllo presidenziale. D'ora in poi, però, se volete davvero rispondere a queste osservazioni sempre più penetranti del Presidente della Repubblica, visto che ogni volta non le ascoltate, pensate ai nomi che date ai provvedimenti e ispiratevi a qualcos'altro che non siano i titoli dei film di Lina Wertmüller.

*(PD)*. Signor Presidente, la Camera ha modificato il testo del decreto uscito dal Senato in alcuni aspetti in verità del tutto marginali. Faccio qualche esempio. Non si sentiva, io credo, l'esigenza...*(Brusìo).* coloro che non sono interessati ad ascoltare gli interventi, sono pregati di lasciare speditamente l'Aula.

un esempio di correttezza istituzionale da parte dell'Assemblea. Colleghi, chi deve lasciare l'Aula, per cortesia lo faccia speditamente. dicevo, non si sentiva l'esigenza di aumentare il numero dei consiglieri comunali e degli assessori di Roma o delle altri grandi metropoli italiane, ma al Senato la maggioranza e il Governo non avevano resistito alla tentazione di dare questo nuovo impulso alla già ben giustificata campagna di denuncia dell'autoreferenzialità e dei costi eccessivi della politica. La Camera ha invece opportunamente deciso di tornare indietro ed ha eliminato i commi che erano stati inseriti a questo proposito dal Senato.

ad evitare di infilare anche in questo provvedimento norme in materia di abusivismo edilizio e di demolizione di immobili, ma il Governo e la maggioranza hanno evidentemente ritenuto che, fallito nel nulla il noto piano casa, fosse almeno necessario salvare dalle ruspe gli edifici costruiti contro e senza alcun piano. La Camera ha provveduto a correggere

questo provvedimento segna un nuovo passo avanti nel processo di degenerazione del nostro procedimento legislativo. Una

questo potrebbe essere l'ultimo treno prima della fine della legislatura, ed è giusto che siano in molti a poterci salire. un appello che, come abbiamo visto dai lavori del Senato, non è rimasto inascoltato, tanto che oggi, a pasticcio combinato e, come ho ricordato, soltanto marginalmente corretto, la maggioranza, per bocca del relatore Malan, non prova nemmeno a difendere le scelte compiute, ma si rifugia, previo diligente computo dei commi e degli articoli di altri decreti milleproroghe dei Governi di centrosinistra, nella più paradossale delle vie di fuga: «Sì, noi sbagliamo, ma avete sbagliato anche voi prima di noi». Certo, abbiamo sbagliato anche noi, prima di voi. Ma da quando, senatore Malan, la diffusione di un vizio lo trasforma in una virtù? Non avete voi vinto le elezioni, tra le altre ragioni, anche perché avete garantito agli italiani che la maggiore coesione della maggioranza, la vostra, avrebbe consentito di smettere di inseguire con leggi *monstre*, come questa, la più minuta e assurda pretesa dell'ultimo senatore, dell'ultimo gruppetto di questo Senato? Senato? Proprio l'uso di questo argomento difensivo ("Lo avete fatto anche voi") dimostra la profondità della crisi politica che ha investito il leader costituente

siete impegnati a giustificare il vostro confuso agitarvi tra centinaia di norme e normette prive di un disegno coerente con il riferimento alla parte peggiore della nostra esperienza di governo. Andiamo avanti, dicono ora all'unisono Berlusconi e Bossi, consapevoli di non avere più al loro arco, questa è la vera novità di queste settimane, tra le alternative possibili l'arma delle elezioni politiche anticipate. andate avanti, ma così, con provvedimenti di questo tipo. In essi si possono rintracciare, è vero, anche tentativi di affrontare i problemi seri del Paese, tentativi che finiscono con l'approdare a soluzioni come quelle contenute nel testo al nostro esame, cioè con esiti letteralmente paradossali, figli della debolezza politica del Governo e della sua maggioranza. Porto solo due esempi per dimostrare questa tesi. In primo luogo, è chiaro che l'innovazione tecnologica sta producendo l'esigenza di una diversa soluzione delle norme anticoncentrazione nel settore cruciale dell'informazione radiotelevisiva e della carta stampata. Voi tentate di affrontare questo problema, che è un problema reale, e siete riusciti a farlo in modo tale da affidare al Presidente del Consiglio, al Presidente del Consiglio, con atto amministrativo, il compito di affrontare il tema della concentrazione *antitrust* nel settore in cui egli ricopre una posizione dominante. È un vero paradosso!

sulle quali interviene quel modello. Abbiamo tentato - Governi di centrosinistra e Governi di centrodestra - di fornire una soluzione riformista a questo problema. Non se ne è potuto far nulla a causa della demagogia imperante in ogni campo politico. Il risultato è che adesso, improvvisamente, nel decreto milleproroghe voi intervenite, e stabilite che, quando su un territorio si abbatte una calamità naturale, voi immediatamente gli rifilate una stangata fiscale. È una soluzione paradossale, quella prevista nel decreto, che dimostra plasticamente che voi vi rendete conto di quali siano i problemi, che cercate di affrontarli, ma che la crisi politica che vi attanaglia è tale per cui la soluzione è spesso peggiore del male. *(IdV)*. Signor Presidente, signori membri del Governo, colleghi,

e soprattutto presenta gravi profili di incostituzionalità, specie sulle norme salvabanche e salvainteressi dei banchieri. Andate a sanare ancora una volta l'anatocismo, ossia la capitalizzazione degli interessi su un capitale, affinché essi siano a loro volta produttivi di altri interessi. Il calcolo degli interessi in regime di capitalizzazione composta anziché in regime di capitalizzazione semplice determina una crescita esponenziale del debito, una fiorente attività di capitalizzazione, come più di una volta le sezioni unite di Cassazione hanno stabilito. L'articolo 1283 del codice civile vieta un regime di capitalizzazione composta degli interessi, ovvero il pagamento degli interessi su interessi di periodi precedenti, ma nonostante la tutela approntata dal citato articolo, per oltre mezzo secolo nella prassi bancaria italiana hanno trovato applicazione generalizzata nei contratti di apertura di conto corrente le clausole di capitalizzazione trimestrale Dal 1999 la Corte di cassazione ha più volte affermato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale. Per evitare un contrasto tra il lavoro dei giudici e la prassi, il legislatore ha ritenuto opportuno,

norma transitoria. Tale norma è stata poi dichiarata illegittima, per eccesso di delega e conseguente violazione dell'articolo 77 della Costituzione, dalla Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre 2000, n. 425.

del principio dell'irretroattività della legge, per la disparità di trattamento fra soggetti del testo unico bancario e creditori sottoposti all'anatocismo e per il mancato rispetto dell'autonomia dell'indipendenza della magistratura.

Dunque, sono molti i profili di incostituzionalità rispetto a una norma scritta sotto diretta dettatura delle banche. Dopo i rilievi effettuati dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, con i quali questi aveva eccepito l'incostituzionalità del decreto milleproroghe, specie sulle norme salvabanche, estranee alla materia ed infilate di notte per confondere nel buio la vostra vergogna, milioni di consumatori vessati, usurati e taglieggiati dalle banche avevano confidato in un ravvedimento operoso del Governo e del ministro dell'economia sull'articolo 2-*quinquies*, scritto sotto diretta dettatura del governatore Draghi, dell'ABI e delle banche per far estinguere i diritti degli utenti dei servizi bancari, sanciti ancora una volta da una recentissima sentenza di Cassazione, la n. 24418 del 2 dicembre 2010.

perché in ogni caso la legge non avrebbe mai potuto avere effetto retroattivo sulle migliaia di condanne per anatocismo inflitte dai tribunali agli istituti di credito, a conferma della profezia di Ezra Pound: questo Governo, e la maggioranza che lo sorregge, è il più fedele maggiordomo dei banchieri e dei loro interessi. signori del Governo e della maggioranza, portate sulla coscienza lo svuotamento della *class action*, che non può essere attivata da milioni di risparmiatori truffati ai quali le banche

Non si illudano Draghi, l'ABI, Bankitalia, il ministro Tremonti ed il Governo, che hanno concertato di notte l'ennesimo furto con destrezza a danno dei consumatori, degli enti locali, perché queste pratiche, questa usura legalizzata, praticata per oltre mezzo secolo da un sistema paramafioso, verranno eccepite davanti ai tribunali. «Con usura nessuno ha una solida casa di pietra squadrata e liscia per istoriarne la facciata, con usura non v'è chiesa con affreschi di paradiso (...) con le aureole sbalzate, con usura nessuno vede dei Gonzaga eredi e concubine, non si dipinge per tenersi arte in casa ma per vendere e vendere presto e con profitto, peccato contro natura, il tuo pane sarà staccio vieto arido come carta senza segala né farina di grano duro, usura appesantisce il tratto, falsa i confini, con usura nessuno trova residenza amena. Si priva lo scalpellino della pietra, il tessitore del telaio (...). Usura soffoca il figlio nel ventre, arresta il giovane amante, cede il letto a vecchi decrepiti, si frappone tra giovani sposi, contro natura. Ad Eleusi han portato puttane, carogne crapulano ospiti d'usura». Questa poesia è di Voi, signori del Governo e della maggioranza, siete i fiancheggiatori più fedeli dei banchieri e delle loro pratiche usurarie, che continuano a strozzare le piccole e medie imprese, centellinando gli affidamenti e che, con le loro lungaggini, ritardano la crescita economica per erogare allegri fidi agli Zalesky, Zalesky, agli Zunino e ai loro compari. Sappiate che questo ennesimo decreto salvabanche, che cancella con un colpo di spugna i sacrosanti diritti dei consumatori, frutto di un quarto di secolo di battaglie contro le mafie bancarie, è la dimostrazione più palese dell'usura di un Governo e di una maggioranza, che, per vivacchiare, sono costretti ad andare a braccetto con i banchieri e a ricorrere ai voti di fiducia per tirare a campare senza tirare le cuoia. Voi, signori del Governo della maggioranza, proteggete e sanate le illegalità e, mentre lesinate qualche milione di euro di detrazioni fiscali alle famiglie taglieggiate dalle banche, erogate 141 milioni di euro (solo nel banchieri, per premiare pratiche vessatorie e tecniche usurarie; premiate l'illegalità degli allevatori, sottraendo fondi ai malati terminali; mettete in concorrenza le associazioni di volontariato sul 5 per mille con gli ammalati di sclerosi multipla. Ma anche stavolta, dopo il decreto salvabanche del 1999 e il successivo decreto salvamutui usurari, la Corte costituzionale, che sarà chiamata a pronunciarsi su norme incostituzionali approvate da un Governo fedele servitore dei banchieri, verranno sollevate, nelle udienze già fissate, a partire da lunedì 28 febbraio, eccezioni di incostituzionalità di norme scritte sotto diretta dettatura dei *bankster*, per cancellare 20 anni di battaglie giudiziarie dell'Adusbef a tutela dei diritti di milioni di famiglie. Noi, signori del Governo e della maggioranza, continueremo a tutelare i diritti di milioni di consumatori, delle piccole e medie imprese strozzate e usurate e della povera gente. Voi continuate continuate a difendere gli interessi dei banchieri che continuano a taglieggiare le famiglie. Sarete certamente in buona compagnia.

della nostra storia parlamentare, e in particolare, ancora una volta, dei rapporti tra questo ramo del Parlamento e il Governo. Il senatore Morando ha giustamente ricordato alcuni miglioramenti che si sono avuti

non frequenta le nostre Aule e non parla a Palazzo Chigi: parla in luoghi diversi e svolge la sua attività nei suoi palazzi, di diverso genere - ha dato la colpa al Parlamento.

in una attività importante svolta in Commissione dove abbiamo rivendicato, e in parte ottenuto, la trasparenza del percorso, ma poi abbiamo visto - e ci ha fatto perdere tanto tempo i problemi che ha avuto la maggioranza nei rapporti con il Governo: abbiamo visto senatori utilizzati come portavoce del Governo, nel presentare emendamenti che rispondevano non ad una elaborazione di questa ad esigenze del Governo. Questo ha messo poi il Presidente della Repubblica nelle condizioni di dover rimarcare che non c'era più il tempo, né per l'altra Camera, né per lui stesso, per un intervento di merito. Questo è cosa grave, che ci ha portato ad una situazione di ricatto e ad una cattiva legislazione. A questo proposito, resta aperto il problema della gerarchia delle fonti e degli elementi di delegificazione che restano in questo provvedimento, rispetto non solo al comma 2, di cui abbiamo parlato diverse volte, ma anche alla proroga del Commissario dell'ANSAS e al regolamento che viene istituito su tutto il tema della valutazione, tema che era un punto centrale di questo Governo e su cui si fa tanta propaganda. dicendo che ora il punto non è più che cosa proroghiamo: il punto è perché proroghiamo, e proroghiamo cose che sono oggetto di delega da due anni. Questo lo dico, signor Presidente, colleghi, perché alla domanda «Lei è in grado di governare?» il Presidente *extramoenia* risponde «Non c'è nessun altro che potrebbe governare meglio».

a onor del vero approfitterò di questi pochi minuti per rivolgere sinceri ringraziamenti ai presidenti delle Commissioni riunite 1a e 5a, senatori Vizzini ed Azzollini, nonché a tutti i membri delle Commissioni

proprio non è: immagine che rischia di peggiorare un clima che invece ci deve vedere nei prossimi mesi molto operativi e seri nel confronto sui problemi che dovremo affrontare. Tra l'altro, per quanto riguarda proprio questo milleproroghe, il nostro Gruppo ha presentato poche decine di emendamenti, di cui ne ha discussi meno di una ventina, per cui, alla fine, tutto

Oltre a questo, bisogna anche dire che si è trovata un'intesa ed una soluzione a diversi problemi. Nelle tre settimane e oltre di intenso e ininterrotto lavoro in Commissione, per esempio, si è arrivati all'approvazione di un emendamento identico,

Per esempio si è trovata una buona soluzione per le autorità portuali. Un approfondimento serio con l'opposizione ha portato a limature e miglioramenti delle norme relative al sistema bancario. Questo per dire che non è poi così vero che il Senato, in particolare su questo provvedimento, ha lavorato male e in maniera superficiale. È, a nostro avviso,

Sicuramente avremo la necessità di ritrovarci a lavorare ancora in maniera seria e costruttiva su questi temi, sul piano nazionale delle riforme in particolare, nei prossimi mesi. questo incidente di percorso non faccia passare un'immagine di un Parlamento che non lavora bene, perché è l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno in questo periodo. *(Applausi

signori colleghi senatori, due fiducie in sette giorni! Sembra veramente che il disordine e la mancanza di programmazione sia diventata la regola del Governo. Due fiducie, non per affrontare un'emergenza o per approvare un coraggioso disegno riformatore, o per sciogliere un grande nodo politico, ma per riuscire a far passare il più modesto degli atti parlamentari, quello che, prevedendo decine e decine di proroghe, certifica che o era troppo ambiziosa la volontà del legislatore o è stata troppo debole l'azione del Governo o della struttura amministrativa. Anche in questo caso però non è mancata da parte del Presidente del Consiglio quella attitudine alla menzogna che sembra essere diventata l'orizzonte quotidiano del rapporto con il Paese; menzogne sulle cose grandi e sulle cose piccole, e di fronte al necessario intervento di garanzia del presidente Napolitano ci ha detto appunto, il Presidente del Consiglio, che non era colpa sua: lui si era occupato di un focoso destriero, e scopre di aver creato un ippopotamo. Immagine fantasiosa ed efficace, se avesse qualche parentela con la realtà. Ma il Presidente del Consiglio pensa che di fronte alla nuvola comunicativa in cui noi tutti siamo immersi, di fronte a quei grandi drammi storici a cui assistiamo e che richiederebbero misura e spirito di verità si possa liberamente mentire, si possa attaccare ogni altro organo costituzionale, come ha continuato a fare nei giorni scorsi, si possa dire che perfino la famosa telefonata alla questura di Milano era l'adempimento di un suo preciso dovere, come ci ha detto. questo è il senso del dovere per il Presidente del Consiglio: agire - vedremo se con rispetto della legge o meno - per consegnare una ragazza minorenne, da lui ben conosciuta, avendola a lungo frequentata, ad una prostituta. Direte: che c'entra? Siete ancora fermi come opposizione a queste vicende? Sì, c'entra, perché lo spirito di verità e il senso del dovere è una qualità necessaria della buona politica. Dove stava questo focoso destriero, dunque? È una triste necessità *bipartisan* - certo, *bipartisan* - riconoscere che la volontà la volontà annunciata si è si è tradotta in un fallimento, cioè chi si aspettava il riconoscimento di un diritto non vede soddisfatto quel diritto e penserà che ha fatto male a fidarsi dello Stato. Chi temeva il venir meno di un privilegio si rallegrerà del fatto che il suo privilegio resterà in vigore. Chi, azienda o professionista, si è preparato investendo con risorse umane in tecnologia per affrontare il nuovo quadro normativo, ancora una volta dovrà constatare sconfortato che il suo sforzo di adeguamento è stato inutile. Questo sarebbe, dunque, il focoso destriero descritto agli italiani? Prorogare oltre 60 scadenze per paura che si realizzi un modesto avanzamento? Sì, è vero che anche i Governi di centrosinistra hanno avuto questi problemi, ma nessun Presidente del Consiglio ha avuto il coraggio di definire un focoso destriero l'incapacità di mantenere le promesse fatte agli elettori. Infine, perché è diventato un ippopotamo?

e solo, ancora una volta, l'intervento responsabile ed equilibrato del Presidente della Repubblica ci ha messo una pezza? È stata l'opposizione? È colpa dell'opposizione? No, l'opposizione si è limitata a rimarcare alcune gravi incongruenze, come la questione del cinque per mille e l'insufficienza degli interventi, ad esempio, per le calamità e i terremoti, si è opposta a questa gemmazione di norme estranee. Avevamo ragione: il destriero si è trasformato in un ippopotamo, perché così ha voluto il Governo. Lo stesso Presidente del Consiglio, che se ne lamenta, è l'autore di questa trasformazione: tutto quello che c'è, incluse le nuove tasse, incluse le norme clientelari, incluso il fatto che perfino i teatri dell'opera sono distinti in base all'appartenenza politica delle amministrazioni, compreso il fatto che che si definanziano gli investimenti per la banda larga, infrastruttura tecnologica indispensabile, compreso il fatto che ci si compiace con l'usura, compreso il fatto che si finanziano 72 o 73 evasori fiscali delle quote latte, togliendo i fondi, già molto esigui, al sostegno degli ammalati terminali. Questa è la priorità del Governo: meglio aiutare gli evasori che accompagnare le famiglie di fronte al dramma di assistere i propri cari nella fase terminale della vita. E voi dite di essere il partito della famiglia. Comunque, tutto ciò o è avvenuto per la volontà e l'azione diretta o indiretta del Governo (il nostro meritevole collega senatore Esposito ha firmato come propri decine e decine di emendamenti scritti dalla mano del Governo), oppure è avvenuto per la mancanza di guida politica della maggioranza, incapace di dare una disciplina al delirio emendativo di alcuni suoi componenti. Tutto, comunque, è avvenuto sempre con il parere favorevole del Governo. E questo ippopotamo perciò è nato perché il Presidente del Consiglio lo ha voluto o perché, troppo distratto dai suoi compiti di imputato, non è più in grado di guidare l'azione di governo. Non vedo, dunque, perché si debbano offendere gli ippopotami, animali che nel loro ambiente sono agili e veloci, forti e coraggiosi: non ha, e di cui avrebbe bisogno. Non è un ippopotamo: è una melma fangosa in cui vi siete addentrati senza una bussola e senza una prospettiva che non sia quella della pura sopravvivenza. Per questo vi diciamo: rimettetevi alla volontà degli elettori, che sono in grado di giudicare e di dare finalmente una svolta necessaria per il bene del nostro Paese.

noi dovremmo fare dei decreti di proroga estremamente contenuti, benché il Governo precedente ne abbia fatti di molto più grandi, con finanziarie *colossal*, invece che con una

il ragionamento dicendo che nel 2008 andava bene farlo, salvo poi pentirsene, e dire - nel 2011 - che queste cose non si possono fare. Si è anche detto che noi avremmo vinto le elezioni perché abbiamo promesso di

abolito). Il criterio di valutare la bravura sulla base della brevità delle norme è bizzarro, specialmente da parte di chi ne ha fatte di molto meno contenute di della quantità, vorrei parlare anche della qualità. I nostri elettori - e anche i vostri - avrebbero approvato il fatto che, pur di fare qualche comma di meno, noi non introducessimo in questo provvedimento le norme che, per esempio, sospendono la riscossione delle rate in scadenza per i Comuni terremotati? Avrebbero barattato un comma di meno nel decreto con il far pagare

così,sospendo la seduta. Il senatore Malan è circondato. Senatrice Colli, ci fa lavorare? I membri del Governo possono ascoltare le sedute invece di venire a fare riunioni in Aula?

alle norme che consentono i tempi tecnici per l'accatastamento degli immobili (le cosiddette case fantasma) e alla proroga degli sfratti per un anno

i fondi per gli enti lirici sarebbero stati veicolati secondo preferenze geografiche. Ricordo che ci sono dei criteri oggettivi per indicare gli enti lirici maggiormente efficienti: che poi

difeso sempre quando è finalizzato all'approvazione di norme che servono ai cittadini, e io credo che siano parecchie le norme di questo genere che sono state inserite nel provvedimento, sia nel testo originario sia nei nei numerosi emendamenti che sono stati approvati, il cui numero credo sia una testimonianza del lavoro accurato che, grazie anche ai senatori dell'opposizione, è stato svolto nelle Commissioni riunite, lavoro che ha consentito un esame approfondito degli emendamenti, benché fossero molto numerosi.

alla questione dell'anatocismo e dell'interesse composto anziché dell'interesse semplice. Il senatore Lannutti sa bene che è uno dei grandi temi di definizione dei rapporti. la definizione di questi rapporti debba continuare con sentenze della Corte costituzionale, così come non riteniamo che i cittadini e le imprese e, dall'altra parte, le banche (imprese anch'esse) debbano sempre continuamente risolvere la questione con sentenze e con l'utilizzo del percorso della giustizia civile, che nel nostro Paese ha una tempistica

in tribuna gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Francesco Orioli» di Viterbo. Rivolgiamo a loro il saluto del Senato e gli auguri per la loro attività di studio.

venuto incontro alle richieste di chiarimento nelle Commissioni riunite, provenienti anche dall'opposizione, in particolare in materia di anatocismo e concessioni televisive, ottenendo un voto unanime nelle Commissioni stesse. Ringrazio i Presidenti della 1a e 5a Commissione e tutti i membri delle stesse per il lavoro svolto.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo». La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo». «La

sono contrari alle premesse e favorevoli al dispositivo.

parere favorevole sul dispositivo

ho dato conto di un'interpretazione del Governo sul comma 61 dell'articolo 2 in materia di anatocismo.

Presidente, conosco gli ordini del giorno, ma non ho capito fino in fondo quali sono le proposte alternative dei relatori e del Governo.

blocca-graduatorie e blocca-supplenti, voluta dalla Lega Nord, evidentemente contraddittoria e anticostituzionale, sulla quale molto abbiamo discusso in Commissione prima e in Aula poi, è stata doverosamente eliminata dal Governo nel maxiemendamento approvato alla Camera, a seguito peraltro dell'autorevole intervento del Presidente della Repubblica. Quella norma diceva esattamente che le graduatorie dovevano essere bloccate contempo, diceva che le graduatorie dovevano essere modificate in recepimento della sentenza n. 41 del 7 febbraio 2011 della Corte costituzionale. È chiaro che, compiendo quella scelta, la maggioranza e il Governo avrebbero determinato un caos gigantesco nella gestione delle graduatorie quindi, sull'avvio del nuovo anno scolastico e sul funzionamento dell'intero anno scolastico. Questa scelta, però, era condizionata dalla volontà di prendere del tempo, in attesa di altre e nuove sentenze dei tribunali amministrativi regionali, in attesa di un'altra nuova sentenza della Corte costituzionale, danneggiando gravemente la qualità della scuola pubblica. La norma non vi è più, ma abbiamo bisogno di chiarezza, qui in Parlamento. Quindi, attendiamo che il ministro Gelmini venga molto rapidamente nelle Commissioni competenti e poi in Aula

proporre come verranno definite le nuove norme sul reclutamento del personale docente ed ATA. Sul primo punto, il Partito Democratico fa una proposta e ritengo che questa sia l'unica soluzione possibile per non gettare nel caos la scuola. La proposta consiste nell'approntare, nel prossimo anno scolastico, un piano straordinario di 61.000 assunzioni di docenti e di 38.300 assunzioni corrispondono esattamente i posti vacanti, inclusi i pensionamenti. Si farebbe così un'operazione, non di assunzione di nuove persone, perché quei posti sono già coperti da personale assunto a tempo determinato con una supplenza annuale, ma si farebbe un'operazione di stabilizzazione che finalmente

attuata dal ministro Gelmini. Non si tratta tanto di assunzioni, quanto di immissioni in ruolo e stabilizzazioni. Sulla seconda proposta, quella di carattere generale, ho sentito molti annunci da parte del Governo ma nessuna proposta qui in Aula. Debbo rilevare che è stata assolutamente impropria la scelta del Ministro di di regolare la formazione e in ingresso del personale docente, non collegandola alle modalità di assunzione. È un'anomalia che costituisce un danno e che, per il prossimo anno, determinerà davvero un grande caos nel funzionamento della scuola.

Per la verità, la cancellazione di questa disposizione ha provocato nei senatori campani un'imbarazzata meraviglia, posto che una norma pressoché simile, nell'aprile del 2010, data alla quale faceva riferimento il collega,

maggiore. L'emendamento era dettato quindi da ragioni di equilibrio, dalle ragioni di chi conosce le esigenze e le emergenze di quel territorio e soprattutto da un incauto atteggiamento della Regione Campania, la quale, a seguito dell'approvazione di una norma,

la natura giuridica della laguna veneta non è assolutamente chiara ed è oggetto di contestazione anche in sede giudiziaria da molti e

volto a definire in maniera più chiara la natura, demaniale o privata, o demaniale e privata, delle tre tipologie di area che fanno riferimento alla laguna di Venezia:

la devoluzione a realtà regionali o provinciali del demanio non comporta alcun tipo di conseguenza pratica, perché loro sanno perfettamente

Nel merito, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi in Aula sul tema che riguarda questo ordine del giorno. Come sapete, la Suprema corte di cassazione ha emesso una sentenza importante, direi storica, che riconosce il diritto di tutti i correntisti italiani, siano essi imprese o a vedere rimborsate le somme illecitamente addebitate sui loro conti correnti dal sistema bancario. Come i colleghi ricorderanno, proprio in sede di milleproroghe non abbiamo esitato un minuto a dare il nostro consenso a far sì che fosse introdotta una norma che consentisse alle banche italiane di effettuare operazioni di ripatrimonializzazione in modo da evitare, tra poche settimane, una "strage degli innocenti", cioè dell'intero sistema delle piccole e medie imprese, al momento in cui entrerà in vigore Basilea 3. E quindi abbiamo dato con convinzione il nostro assenso a quella norma che consente al sistema bancario le operazioni di ricapitalizzazione che eviterebbero una tragica stretta creditizia sull'intero sistema produttivo italiano. Ciò detto, però, concedere una mano per affrontare un problema di sistema-Italia non significa dover tacere su chi tenta di prendersi l'intero braccio. specifica norma prende l'intero braccio, perché significa contraddire una sentenza della Corte di cassazione che consente a tutti i correntisti di riavere il maltolto da parte del sistema bancario sui loro conti correnti: far partire la prescrizione decennale dal momento in cui si chiude il conto corrente significa in realtà azzerare tutti i contenziosi fino all'anno 2000 (è il tema che viene definito con il nome più noto di anatocismo). Noi non vogliamo ovviamente mettere nessun intralcio a questo milleproroghe che scade domani, e non abbiamo fatto emendamenti su questo argomento. Si accolga però almeno un ordine del giorno che impegni il Governo a provvedere nei tempi futuri, nelle prossime settimane, a sanare questo *vulnus* che riguarda milioni e milioni di cittadini italiani, lesi nel loro diritto ad essere rimborsati laddove si dimostri, come tanti contenziosi in atto stanno dimostrando, che hanno il sacrosanto diritto di ricevere dalle banche i soldi indietro laddove quei soldi sono stati addebitati ai conti correnti in un modo illecito. Questo è l'ordine del giorno G119. Capisco che il sabato mattina non favorisce l'attenzione su questo punto, ma vi prego, signori colleghi, di fare attenzione, perché è un semplice ordine del giorno non modifica in nulla l'*iter* del decreto, ma dà un segnale di speranza alle famiglie, agli individui, alle piccole e medie imprese e al sistema economico-produttivo italiano nel ribadire che i diritti in questo Stato vengono mantenuti mantenuti e la possibilità che, laddove vengano riconosciuti, chi ha sottratto illecitamente fondi dai conti correnti sia obbligato a restituirli. Se non passa neanche un ordine del giorno del genere, significa che stiamo sancendo (ciò è scritto nel decreto) che tutto ciò che è avvenuto negli ultimi venti anni in Italia, con la prevaricazione del sistema bancario sui correntisti - prevaricazione

dei cittadini mi sembra esagerato. Essendo un ordine del giorno, mi richiamo all'ovvia responsabilità di tutti i colleghi perché quest'Aula possa dare un segnale di speranza ai cittadini italiani sul fatto

(articolo 2935 del codice civile) che va letta in riferimento alla decadenza dei diritti nascenti dalla mancata contestazione: nei

bancario). Ripeto: abbiamo una dimestichezza con queste materie, perché siamo stati i protagonisti anche dell'udienza

diamo 141 milioni di euro per mettere a posto i conti, ma chi pensa ai problemi e ai diritti della povera gente, dei consumatori, delle piccole e medie imprese? Quindi, noi Quindi, noi dell'Italia dei Valori voteremo a favore.

di poter far fare ingresso nel provvedimento alla norma chiamata salva-banche (quella cioè di patrimonializzazione delle banche per mezzo del riconoscimento di uno speciale credito di imposta), fornimmo il nostro assenso a condizione che venissero stralciate due norme: la norma che disciplinava in modo alquanto discutibile

cittadini, famiglie e imprese. Il Governo preferì tirare diritto, e la maggioranza votò quella norma, così come era stata proposta dal Governo.

spero che il Governo lo voglia assumere in quest'Aula, approvando questo ordine del giorno e i successivi ordini del giorno, tra cui uno del nostro Gruppo, a prima firma del senatore Barbolini, di cui chiederemo ugualmente la votazione. sarà certamente travolta dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, poiché affida l'esercizio di un diritto - quello alla restituzione di interessi illegittimamente percepiti dalle banche al tempo dell'esercizio dell'azione civile. In altre parole, i cittadini che hanno già esercitato questa azione e hanno ottenuto la restituzione vedono salvaguardati i loro diritti; coloro che hanno un giudizio in corso, o che addirittura hanno avuto una sentenza di primo o di secondo grado favorevole, invece soppresso il diritto alla restituzione. È una norma, quindi, che non resisterà al vaglio della Corte costituzionale e che è urgente

sull'ordine del giorno G200 del senatore Battaglia, che accoglie gli argomenti che sono stati formulati.

Signora Presidente, sull'obiettivo di fondo vi è - lo posso constatare dalle conversazioni che stiamo avendo con i colleghi - una larga convergenza e una diffusissima sensibilità. Aggiungo che, dal punto di vista procedurale, ove dovessimo trincerarci dietro la forma e dire che l'ordine del giorno semplicemente va a contraddire la norma del testo, mi dovrei chiedere allora perché sia stato dichiarato ammissibile l'uno o l'altro.

che non complichi i problemi, ma li risolva, e mi pare largamente nel senso che gli onorevoli presentatori di questi emendamenti stanno auspicando. Se così è, e riconosciamo che l'interesse di fondo da tutelare (che è quello dei risparmiatori, degli operatori economici, e non certo il privilegio di chicchessia, nemmeno degli istituti di credito) deve essere tutelato, dico - mi permetto di dire - che se, come ho ascoltato, i relatori sono intenzionati a proporre una qualche riformulazione che renda meno drastico il senso dei testi, ma che ci permette di affermare il principio in prospettiva, non debbo suggerire niente, ma direi ai presentatori degli emendamenti

(non è questa la sede, e stiamo, in questo senso, abusando di tale strumento, ne convengo), possiamo però affermare, forse all'unanimità, un principio. Quindi faccio un appello perché, recependo i segnali positivi che vengono sia dal Governo, che dai relatori,

possano ottenere confluenze più ampie sull'argomento, nella sostanza.

l'ordine del giorno G200, così com'è, attiene, con tutto il rispetto per le opinioni del senatore Battaglia, all'interpretazione della norma, norma, come ha detto giustamente il collega Baldassarri. Si dice: facciamo in modo che la norma venga interpretata dai magistrati nel modo meno dannoso possibile, il che è impossibile, perché la norma è chiarissima.

altrimenti è un atteggiamento ipocrita - chiedo scusa - perché non si può interpretare una norma di legge chiara in modo difforme dalla lettera della norma.

a difendere questo principio con la presentazione dell'ordine del giorno G200, siamo d'accordo su quanto si è detto e convergiamo sull'ordine del giorno del senatore Battaglia, che verrà subito dopo votato.

fa capolino e finisce per confondere le idee. In questo provvedimento c'è una norma importante che rende omogeneo un regime fiscale adottato nei confronti delle banche rispetto al regime in uso negli altri Paesi europei. Per questo siamo tutti d'accordo, e anche le opposizioni hanno manifestato interesse a che venisse inserita

totalmente ostile ai consumatori e che contiene una palese ingiustizia, immotivata e ingiustificata, che distorce il senso di una sentenza della Cassazione:

perché basta leggere il testo in italiano dello stesso per capire che è l'ennesima presa in giro dei cittadini italiani, soprattutto dopo il voto contrario sul precedente ordine del giorno

la volontà del Governo si esprime nelle Aule parlamentari - e di questo i parlamentari devono tener conto - e non attraverso interviste giornalistiche,

i consumatori, i cittadini, le famiglie e la povera gente sapranno chi ringraziare: continuate ad andare a braccetto con i *bankster* che hanno ridotto sul lastrico le famiglie.

Senato e Camera; quindi, da questo punto di vista, l'emendamento potrebbe essere ammissibile. Mi si dice peraltro da parte degli Uffici che c'è una questione di inammissibilità. Vorrei spiegare la ragione, prima di dare una conclusione sul punto, per cui abbiamo presentato questo emendamento. Stiamo assistendo ad un aumento dei reati in materia di corruzione, che è stato messo in luce tragicamente dal procuratore generale della Corte dei conti e dal presidente della Corte dei conti, già presidente dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici e sugli appalti pubblici. Il presidente Giampaolino, in particolare,

Il problema della corruzione in questo Paese è serissimo, ma a fronte della necessità di combatterla il Governo si muove in senso assolutamente contrario:

noi dobbiamo necessariamente insistere per riportare l'attenzione sulle norme anticorruzione. Peraltro, se l'emendamento viene ritenuto inammissibile e siccome immagino che il provvedimento milleproroghe dovrà essere approvato nella giornata, anche contro la nostra volontà, ritiro

Presidente, per la verità in Commissione

chiedo scusa. Effettivamente, non c'è alcuna ragione per la quale tale norma sia stata cassata alla Camera. Si tratta tecnicamente di una proroga, e la ragione è semplicissima:

accolgo l'invito alla sua trasformazione in ordine del giorno, nello stesso testo approvato in Commissione.

perché tratta uno degli argomenti più delicati di questo complesso e pasticciato provvedimento. Noi rischiamo due cose: che il 1° aprile non vi sia più alcuna normativa *antitrust* sul tema dell'incrocio stampa‑televisione, una vicenda unica nel suo genere, ossia che il Presidente del Consiglio, che è diretto interessato, può prorogare con suo decreto forma di *antitrust* residuale fino a fine anno. È vero che è stato accolto un ordine del giorno, ma siccome ho visto con grande piacere una dichiarazione positiva anche del senatore Gasparri, mi chiedo allora perché non approvare questo emendamento, che è chiaro, netto, inequivoco ed evita qualsiasi *vacatio legis*. siccome la questione è molto importante, vorrei ricordare al senatore Vita che, d'intesa con il Governo e nel testo varato dal Senato, con tutte le solennità dei lavori che hanno accompagnato il decreto milleproroghe, era stata modificata la legge Gasparri che prevedeva un limite temporale al divieto di incroci, cioè alla possibilità da parte dei giornali di comprare televisioni e viceversa.

del Senato avevano varato. Quindi, noi siamo favorevoli a protrarre quel termine. Se oggi ci si limita all'ordine del giorno e non a una modifica del testo legislativo, non è colpa del Senato, che quella modifica aveva fatto con legge, e che poi qualcun altro ha chiesto di modificare, non certamente noi.

Signora Presidente, ancora una volta invito, anche se è un'esortazione vana, che cadrà nel vuoto, a riflettere sui danni che verranno inferti a milioni di consumatori e di piccole e medie imprese da questa norma salvabanche. Il nostro emendamento tendeva a salvare i diritti

stati "sparati" per indurre la maggioranza a fare quadrato. Sono molto meno e, se vi fosse stata la *class action*, forse si poteva arrivare a quella somma. Ma la *class action* non c'è,

di compromesso, cioè di applicare il nuovo termine di prescrizione solo per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore di questa legge, facendo salve non soltanto le somme rimborsate e le sentenze passate in giudicato ma anche i giudizi pendenti. Io sono personalmente assolutamente convinto che questa sarà alla fine la soluzione che sarà sancita

Presidente, nell'ipotesi di trasformazione in ordine del giorno sei senatori, i cui nomi ho fatto prima, sarebbero favorevoli.

si è così concluso l'esame degli emendamenti. Poiché le dichiarazioni di voto si svolgeranno in diretta televisiva, al fine di consentire la predisposizione dei necessari adempimenti tecnici, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 14.

continua a veder cadere uno dietro all'altro, come birilli, drammaticamente, una serie di dittatori amici, fa raggiungere alla pressione fiscale il valore massimo degli ultimi 15 anni. anni. Fuori di qui, i nostri concittadini fanno i conti con i prezzi dei carburanti schizzati alle stelle: anche il prezzo della benzina raggiunge un record*.* Non è male per il Governo Berlusconi, per l'uomo che era sceso in politica con lo slogan «Meno tasse per tutti». Oggi torna in quest'Aula un decreto che abbiamo già esaminato, e sul quale già ci siamo espressi con un voto di fiducia, perché il presidente Napolitano ha richiamato il Parlamento e il Governo ai propri doveri. In realtà, in questi giorni l'aveva già fatto l'opposizione nel suo complesso, dicendo dicendo che il decreto si era trasformato in una sorta di finanziaria, in una sorta di carro sul quale erano saliti piccoli e grandi favori. Il Presidente della Repubblica, al quale, signora Presidente dell'Assemblea, esprimo il mio rispettoso ringraziamento, ha richiamato tutti al proprio dovere. Potevamo farlo direttamente noi, potevate farlo direttamente voi. Non l'avete fatto e quindi siamo qui a votare il decreto milleproroghe. Vi sono tanti motivi per esprimere un voto contrario, e proverò ad elencarne alcuni. È sinceramente scandaloso che, per premiare un po' di furbetti amici della Lega Nord, sulle quote latte si siano presi i soldi dal fondo per le cure ai malati di cancro.

se prima avvertivamo poco la sua presenza, adesso l'avvertiamo ancora meno. Il FUS fu lasciato dal Governo Prodi con una dotazione intorno ai 500 milioni di euro e oggi sono 250. Abbiamo chiesto più volte di rafforzarlo. La cultura, lo spettacolo sono uno dei grandi momenti di lavoro, di investimento, di stimolo turistico per il nostro Paese. Ebbene, voi avete scelto di non finanziarla. Avete dato un po' di soldi alle strutture, alle fondazioni liriche, scegliendo anche in questo caso chi premiare e chi no: quelle amiche della Lega, Milano e Verona, lasciando il resto ai margini.

assumendo giovani architetti, tecnici, cercando di far crescere la tutela. State smantellando la tutela della cultura del nostro Paese, con quello che ne conseguirà. Non è solo il problema

voglio dire che abbiamo di fronte a noi un decreto cresciuto spropositatamente nei vari rimaneggiamenti, nel tentativo di accontentare tutti i pezzetti della vostra maggioranza raccogliticcia. Siamo passati da 25 a 196 commi, fatti di piccoli e grandi prebende: mance, appunto, per quel complesso di interessi che tiene insieme la vostra maggioranza. Per questo e per tanti altri motivi, voteremo contro questo decreto, che offende le istituzioni, mette le mani nelle tasche degli italiani (l'euro sul cinema), segna un altro triste momento della lunga agonia della maggioranza e del Governo, non più in grado di governare. Prima si chiuderà questa pagina, meglio sarà per l'Italia. Signora Presidente, l'Italia dei Valori conferma per la seconda volta in Senato il suo voto contrario a questo decreto-legge che si è rivelato, rispetto ai bisogni, alle necessità della nostra gente, per quello che realmente è. E' un contenitore vuoto di mille prese in giro e di mille ipocrisie. E la prima vergognosa ipocrisia - lo dico al Ministro, al rappresentante del Governo - è quella del Presidente del Consiglio, che a cose fatte ha fatto finta di non sapere nulla e ha disconosciuto il provvedimento, senza minimamente preoccuparsi che, così facendo, ha disconosciuto la sua stessa maggioranza, che ha prodotto ben quattro quinti degli emendamenti rispetto alla versione originaria. La seconda ipocrisia è quella del ministro Tremonti che, dopo aver fatto consumare giorni interi per avallare coperture economiche a queste o a quelle proposte emendative, ha assunto il ruolo di salvatore della Patria tagliando quello che voleva e, comunque, meno di quello che avrebbe dovuto, secondo le vere indicazioni del Capo dello Stato. Allora, sono iniziate le sforbiciate. Cerchiamo di capire come sono avvenute. Via la proroga del blocco alle demolizioni delle case abusive in Campania, via la proroga delle concessioni per gli operatori danneggiati dall'eruzione dell'Etna. Non importa poi se c'è lo scontento dei parlamentari del Sud: tanto a loro si dirà che si farà il piano per il Sud. Si taglia lo slittamento delle graduatorie territoriali e provinciali, tanto richiesto dalla Lega. Non importa se poi la Lega è scontenta, perché il loro scontento verrà compensato dalla proroga delle multe dei truffatori delle quote latte. Scompare inoltre la possibilità per i Comuni di oltre un milione di abitanti di aumentare il numero degli assessori: non importa se il sindaco Alemanno si è infuriato e ha minacciato che non finisce qui. Ed allora, che cosa lascia veramente il Ministro dell'economia, così attento alla ricerca degli equilibri del bilancio dello Stato? Lascia la brutta sorpresa per i cittadini sull'anatocismo degli interessi bancari, bancari, le norme fiscali sulla deducibilità delle perdite delle banche, la revisione della tassazione dei fondi comuni, la proroga delle vendite delle quote determinate in eccesso per le banche popolari. Banche, banche, banche! Un bel regalo, non c'è che dire! E già che c'è, questa maggioranza, visto che non si sa mai che cosa può accadere in futuro, introduce la cancellazione al 31 marzo del divieto di acquisto di giornali da parte di proprietari di gruppi televisivi, in modo da aprire, a partire dal 1° aprile, la possibilità di uno *shopping* della carta stampata da parte di Mediaset e del suo proprietario,

è quella consumata ai danni dei lavoratori, delle famiglie, delle imprese e dei piccoli artigiani, a cui era stato fatto credere che questo provvedimento, per via del titolo ambizioso che gli era stato dato, avrebbe contenuto misure e interventi a loro sostegno. cosa ha pensato bene di fare questo Governo per le famiglie, dopo che aveva promesso il quoziente familiare e il fattore famiglia? Ha pensato di aumentare le tasse: dopo la tassa di soggiorno, la tassa di scopo e le addizionali IRPEF introdotte con il federalismo municipale, con questo decreto consentite e approvate la tassa sul cinema, sui rifiuti, sulle energie e addirittura sulle disgrazie, perché le Regioni, se saranno colpite da calamità, dovranno aumentare le tasse. Alle imprese voi dite che occorrono 93 milioni di euro per coprire il decreto milleproroghe. Queste risorse dove le prendete? Le prendete dalle compensazioni dei crediti d'imposta, che dovevano essere dati alle imprese e saranno pagati un anno dopo, se tutto va bene e se nel frattempo le imprese non avranno chiuso i cancelli. Per non parlare dei lavoratori precari, alla cui tutela sociale non è stato destinato un solo euro di risorse aggiuntive. Altro che appello ai principi della Costituzione! Voi, signori rappresentanti del Governo, avete bisogno di un appello alla decenza, perché mentre avveniva tutto questo avete proposto in contemporanea un bel regalo al sistema dei partiti con la sanatoria per chi era in ritardo nella richiesta di rimborso elettorale, un colpo di spugna alle multe per le liste appese in maniera abusiva dei manifesti e il ripristino dei gettoni di presenza per i consiglieri di circoscrizione. Onorevoli colleghi, abbiamo tutti apprezzato e rispettato le parole e i contenuti della lettera che il Capo dello Stato ha inviato ai Presidenti di Camera e Senato. Al Presidente della Repubblica spetta il compito, che assolve con autorevolezza, di un richiamo imparziale al rispetto dei principi sanciti dalla nostra Costituzione. A noi parlamentari, però, e soprattutto a noi parlamentari dell'opposizione, spetta il compito di far capire fino in fondo che cosa sta realmente accadendo nel nostro Paese e in questo Parlamento, perché sia chiaro l'uso e l'abuso della decretazione d'urgenza che ha distinto l'azione di questo Governo. Non si tratta infatti - come si vuol far credere in questi giorni - dell'esigenza di un decisionismo moderno, europeo ed efficiente che deve dare risposte tempestive alle difficoltà del nostro Paese, ma solo dell'espressione di una mentalità ideologica distorta che ha pervaso questo centrodestra e fa credere a Berlusconi di essere il padrone dell'azienda Italia e, in un delirio di onnipotenza, di poter decidere lui dove finisce l'arbitrio e dove inizia la legge. Per questo il Parlamento è soltanto una perdita di tempo, un ingombro e un fastidio. Per altro verso, la proliferazione e la diversità delle norme e delle materie trattate, che hanno portato questo decreto a gonfiarsi come un *soufflé*, passando dai 25 commi iniziali ai 196 della prima lettura, e dove si è inserito di tutto e di più (dagli operatori del salvamento acquatico al numero degli assessori di Roma) nasconde un problema ben più grave, che è il problema dei problemi: dei problemi: che tutto questo serve soltanto a mascherare l'assenza di un progetto credibile per il nostro Paese e di una visione d'insieme delle priorità e dei bisogni, e mette a nudo le contraddizioni di una maggioranza appiccicaticcia che vive alle giornata, non «aspettando Godot», aspettando la pensione, che viene tenuta insieme con qualche contentino, con le mance e con l'illusione che distribuire contributi a fondazioni amiche o difendere gli interessi di banche e fondi di investimento possa aiutarla a conservare un minimo residuo di contatto con il Paese. Alcune settimane fa il Governo ha fatto finta di accorgersi che bisogna finalmente fare qualcosa per la crescita del nostro Paese. Ha annunciato l'ennesimo piano per la crescita, non una scossa all'economia, come ha detto. È stata una mossa da *cabaret.* è una vergogna constatare l'inconsistenza vuota di quei provvedimenti e la stupefacente faccia tosta con cui sono stati presentati per l'ennesima volta,

è un piano aggiornato, modificato, ritoccato, ripresentato e mai attuato. Per la riforma fiscale, che doveva essere la vera riforma epocale e che veniva data per approvata entro il 2010, non siete stati neppure in grado di modificare minimamente l'IRAP, che con questo provvedimento resta così come è, con un'ennesima proroga. A questo Governo, fermo e assediato dalla sua stessa maggioranza (lo abbiamo visto in questo decreto) lasci dire, signor Ministro, anche vedendo i Ministri e i Sottosegretari che si dimettono - dalle inchieste giudiziarie, noi non chiediamo di risolvere i problemi del nostro Paese. Potevate farlo: avevate i numeri e non siete stati capaci di farlo. di farlo. Come italiani, vi chiediamo, però, di restituirci credibilità, perché siamo stanchi del fatto, che all'estero, per le politiche del cucù e del baciamano dei dittatori, stanno ridendo di noi. vi chiediamo di restituirci dignità, perché il 6 aprile le telecamere di tutto il mondo assisteranno al processo all'imputato Berlusconi, dove sfileranno, una dopo l'altra, ballerine, attricette e giocolieri. *(Applausi dal di restituire alle istituzioni onore, nel rispetto dell'articolo 54 della Costituzione della nostra Repubblica. Vi è un solo modo per riavere tutto questo: restituire ai cittadini il diritto alla loro sovranità.

affronterò il tema di questo provvedimento da un punto di vista preciso, quello di un provvedimento emblematico del rapporto malato che vi è tra il Governo - questo Esecutivo - e l'istituzione parlamentare. parlamentare. Nella sua cultura di riferimento - se di cultura si tratta, ma comunque nella sua prassi operativa, nel senso che ispira la sua azione - questo Governo non considera il Parlamento l'interlocutore naturale e privilegiato per la definizione dei provvedimenti legislativi nell'interesse generale: lo considera un fastidio, un problema, una difficoltà da bypassare, in qualche caso un luogo da conquistare o, forse, meglio, da adescare. Mi pare che le cronache di questi giorni ce lo dimostrino: questa continua conta di parlamentari, questo ascrivere l'ultimo successo alla maggioranza nella capacità di captare le incertezze, la necessità di sostenere un Esecutivo precario, debole e incerto di fronte all'opinione pubblica e nella sua azione di governo attraverso il puntello di un Parlamento fragile, soprattutto per la sua modalità costitutiva. Il Parlamento è in queste condizioni di fragilità, nella sua dignità, per come esso è costituito, per una legge elettorale inaccettabile, che induce nelle peggiori tentazioni ogni *leadership* di partito. L'attuale legge elettorale, infatti, tira fuori il peggio della politica: le cronache hanno confermato in modo imbarazzante come è fatto questo Parlamento e quali sono le reali motivazioni che assistono l'azione politica. Dentro questo c'è poi una prassi operativa: decreti‑legge più fiducia; provvedimenti come il milleproroghe che partono per perseguite alcune finalità e diventano il contenitore *omnibus* di ogni risposta ai tanti contraenti di questa maggioranza (contraenti piccoli e grandi, ognuno con la propria questione da affrontare). Il provvedimento diventa inaccettabile, indigeribile e incontra la doverosa, ma essenziale, funzione arbitrale del Capo dello Stato, che riconsegna al Parlamento, se lo vuole cogliere, un momento di dignità nel riappropriarsi della sua funzione. di questa contrattazione, inoltre, sono contenute vicende emblematiche dello stato dei rapporti di questa maggioranza. Ci sono contraenti deboli, piccoli, con alcune micragnose esigenze, e contraenti forti, come la Lega, che è il vero azionista di riferimento, il vero tutore, il cui profilo incombe su questa maggioranza ed impone scelte fondamentali, come il federalismo, che è irricevibile nella sua forma, non soltanto proceduralmente come disse il Capo dello Stato legislativo che il Consiglio dei ministri varò dopo la bocciatura della Commissione bicamerale. È irricevibile nei suoi contenuti essenziali, per l'aggravio fiscale e perché non si fa carico delle esigenze di perequazione e di equità che erano contenute nella legge delega.

C'è una misura che non deve essere superata quando si affronta con determinazione la rappresentanza, e la misura è il senso dell'interesse generale. Voi, con questa tutela esasperata degli interessi di un territorio, rischiate di varcare quella misura.

anticipando un partita difficilissima, dato che questo Esecutivo ci ha già preannunciato interventi radicali in materia di giustizia, con modifiche anche di rango costituzionale. La vigilanza, il baluardo del Capo dello Stato, sarà una misura di garanzia per tutti, per evitare che attorno a quella partita vengano stravolte le regole alla nostra

secondo cui molte disposizioni aggiunte in sede di conversione sono estranee all'oggetto, quando non alla stessa materia, del decreto-legge. anche provato a dire che, così facendo, veniva meno l'elemento che dovrebbe essere sempre contenuto in un dispositivo normativo, cioè la pedagogia delle leggi. Inoltre, ancora il Presidente della Repubblica scrive: non mancherebbero spazi, attraverso una leale collaborazione tra Governo e Parlamento, da un lato, e fra maggioranza ed opposizione, dall'altro, per evitare che un decreto-legge concernente essenzialmente la proroga di alcuni termini si trasformi sostanzialmente in una sorta di nuova legge finanziaria dai contenuti più disparati.

né in Germania, né in Francia, né in Inghilterra, dove le leggi si fanno e poi si applicano) che contiene certi elementi è stato trasformato in un carrozzone, dove davvero difficile immaginare potesse stare tutto e quasi il contrario di quel tutto, così come è poi avvenuto.

per poi adottare decisioni necessarie con altri interventi. Non è stato così: è stato fatto un po' di *restyling*; è stata cancellata qualche scritta troppo vistosa e si è rimesso il carrozzone in strada. Su

Insieme ci sono i provvedimenti per Poste italiane, che può acquistare pacchetti delle banche per diventare essa stessa una banca. messa in discussione di un fondo di 100 milioni di euro, che era stato previsto nella legge di stabilità per affrontare i gravi problemi di malati di e la possibilità di prorogare i termini per il pagamento delle multe per chi era stato sanzionato. Non vi pare che questo coincida in qualche modo con uno sganciamento delle regole dai comportamenti? Non è come dire di voler aiutare gli ultimi e chiudere gli occhi sui primi, intesi come i più furbi di turno? Mi pare francamente che ci sia buon motivo per dire che questo non è un buon provvedimento. Qualcuno mi ha suggerito che ci sono 90 milioni di euro per la mia Liguria dovrei tenerne conto. Ne tengo conto, e ringrazio per questo atteggiamento intelligente. Penso che non si dovesse aspettare il milleproroghe,

Mi pare che si faccia riferimento ad una leva fiscale, ancora una volta impropria, ancora una volta inopportuna. «Il carrozzone va avanti da sé» scrive un noto cantautore romano e, quindi, non avete bisogno certamente di noi. Capita ‑ ultimamente è capitato spesso in questo Paese ‑ che le parole e i colori vengano sequestrati un po' da una parte: capita al verde, all'azzurro, al viola e perfino agli *slogan* durante le partite di calcio. e diventa difficile usarlo per altro. Stava per capitare anche alla parola responsabilità: poi, forse, c'è stato un ripensamento, e forse

questa mattina coincide esattamente con un voto contrario a questo provvedimento, per non essere chiamato domani a correità nel pensare ad un'Italia in questo modo, perché noi la pensiamo davvero diversamente. *(FLI)*. Signor Presidente, noi avevamo già votato contro il provvedimento milleproroghe per quello che è diventato in questi anni e, nello specifico, per quello che è in questa occasione. Poi, i noti eventi hanno portato ad un ulteriore passaggio in quest'Aula. Anche a nome dei sei senatori dell'ex Gruppo Futuro e Libertà per l'Italia, l'Italia, quello che abbiamo visto e vissuto questa mattina in quest'Aula ci conferma ancora di più in questa determinazione. Nello specifico, per non tediare i colleghi, in un argomento rilevante che riguarda milioni e milioni di cittadini, di famiglie e imprese,

però, avevamo sollevato, con un ordine del giorno, un problema che mi sembrava largamente condiviso in tutta l'Aula, anche se solo in apparenza. Infatti, nel momento in cui si fa chiarezza sulla necessità di sanare un *vulnus* inaccettabile,

danneggiato o che comunque si è visto sottrarre somme di denaro attraverso i conti correnti bancari, ha subito sottrazioni illecite,

Non c'entra nulla il problema della stabilità del sistema bancario: su quel punto avevamo dato e continuiamo a dare il nostro sostegno per dare forza di patrimonializzazione al nostro sistema bancario ed evitare

non si può dire di essere contrari al principio, perché sarebbe dirompente in termini di opinione pubblica, quindi si dice di essere favorevoli a quel principio, ma poi nel voto concreto dell'Aula parlamentare

addurre come argomento che in un articolo di stampa il Ministro dell'economia si sarebbe impegnato nei prossimi giorni ad affrontare il problema. Mi pare che dal punto di vista della correttezza istituzionale questo sia

maggioranza di quest'Aula, che riconosce ai cittadini italiani il diritto sacrosanto di vedersi rimborsare le somme illecitamente sottratte attraverso

siamo in presenza, dopo una crisi economica mondiale, di una nuova crisi internazionale di proporzioni importanti - lo vedete tutti - che rischia di tradursi in una crisi umanitaria con milioni di profughi, milioni di poveracci che vengono spinti dalla fame e dalle guerre a cercare un altro posto. In apertura vorrei quindi rivolgere il pensiero del Gruppo della Lega ai flussi degli immigrati che stanno scappando dalla Libia e dal Nord Africa. Questa drammatica vicenda non può ricadere solo sulle spalle del nostro Paese. Di fianco a questi, vi sono migliaia di europei e nostri connazionali che cercano di rientrare in patria. Su questo punto vorrei ritornare. Oggi esaminiamo un provvedimento che concretamente pone mano ad alcuni problemi: a volte, problemi che possono sembrare piccoli, ma sempre problemi molto reali sono, e che toccano i nostri cittadini, le nostre famiglie ed imprese. È su fatti concreti che verremo misurati, e che siamo misurati dai nostri cittadini. È questo un provvedimento che aiuta la nostra economia, mantiene centinaia di posti di lavoro, in un momento di grande difficoltà e in un momento in cui abbiamo bisogno di compattezza: fatti concreti che sono contenuti in questo decreto, per merito anche del nostro lavoro (abbiamo presentato in prima lettura del provvedimento solo pochi e mirati emendamenti, circa 90, per cento di quelli che sono stati presentati, in gran parte dell'opposizione, dimostrando che vale la qualità e non la quantità, e si evitano anche così sprechi). Ad esempio, gli interventi sulla navigazione sul lago Maggiore, sui laghi di Garda e di Como, che devono funzionare, e c'è bisogno di soldi. Rifinanziamo gli enti lirici di Milano e di Verona, nonché l'orchestra sinfonica «Giuseppe Verdi», che sono istituti culturali famosi, che rendono orgogliosi gli italiani nel mondo. C'è il rispetto della promessa del presidente Berlusconi e del ministro Bossi agli alluvionati del Veneto e ad altri alluvionati, ad esempio quelli della Liguria, con nuovi finanziamenti; ci sono misure che danno una mano sul Patto di stabilità agli enti locali. E poi c'è una norma che incide su quei piccoli Comuni montani, come quelli del mio territorio, che confinano con le Province autonome di Trento e di Bolzano e che hanno bisogno di un intervento puntuale. Siamo molto legati a questo provvedimento voluto dal ministro Calderoli. Ci sono insomma fatti concreti che interessano le comunità locali, interessano le persone coinvolte, interessano chi vive e lavora nel nostro Paese: per esempio, noi evitiamo che i lavoratori che hanno cause presso la Corte di cassazione debbano pagare e siano vessati da un contributo che difficilmente riuscirebbero a pagare. C'è, inoltre, il fondo del 5 per mille che viene dato alle associazioni di volontariato: e, queste sì, sono una risorsa fondamentale per tutto il nostro Paese. Sempre nel segno dell'aiuto, condividiamo le misure di sostegno per il sisma dell'Aquila e dell'Abruzzo. Vorrei qui ricordare la solidarietà di tante associazioni e persone che anche dalle nostre Regioni del Nord sono andate per prestare il loro contributo. Ci sarebbe poi da parlare degli interventi sul sistema bancario per mettere in sicurezza le banche dagli attacchi finanziari, e quindi per garantire il risparmio delle famiglie e per assicurare il credito alle imprese, come pure di tanti altri argomenti. Mi rivolgo quindi all'opposizione per chiedere: chiamate poco o inutile tutto questo? Molte sono poi anche le misure a favore e a riconoscimento del lavoro degli operatori delle forze dell'ordine e della sicurezza, a beneficio dei cittadini. I casi degli sbarchi in questi giorni sono emblematici, e ringraziamo il ministro Maroni per il pronto intervento. Riprendendo quindi il dramma ricordato all'inizio, bisogna dire che l'ostilità dei Paesi nordeuropei, contrari a dare aiuti e a partecipare alla gestione dei flussi degli immigrati che stanno fuggendo dalla Libia e dai Paesi del Nord Africa, è vergognosa. È ora che chi ha sempre difeso questo modello di Europa apra gli occhi. È inaccettabile che l'Europa difenda solo gli interessi delle grandi banche e della finanza e si tiri indietro di fronte a un'emergenza umanitaria di queste proporzioni. Lega Nord ha presentato una mozione al Senato per dare mandato al nostro Governo di pretendere, da parte di tutti i Paesi dell'Unione europea, un forte impegno e una politica comune in tema di immigrazione e asilo. Siamo quindi pienamente soddisfatti per quanto fatto e ottenuto, nel segno della fiducia che i cittadini-elettori ci hanno dato ed alla quale rispondiamo con concretezza e ottenendo rinnovato sostegno. Questo Paese si cambia lavorando, e non facendo continue polemiche. Esiste una maggioranza, e non è vero, come dite voi dell'opposizione, che il Governo non è in grado di governare: esso è in grado di governare e lo dimostriamo coi fatti. C'è una maggioranza che va avanti con convinzione. Crediamo che questo Paese di tutto abbia bisogno tranne che di calunnie, polemiche e risse infinite. Ci interessano le leggi che discutiamo ed approviamo, e non siamo e non ci sentiamo assolutamente indeboliti come qualcuno vorrebbe. Oggi, ad esempio, mostriamo come in quarantott'ore, con serenità, abbiamo accolto alcune modifiche che legittimamente il capo dello Stato Napolitano ha raccomandato. della nostra capacità ricordiamo il grandissimo e storico risultato ottenuto in quest'Aula, mercoledì 23 scorso, con l'approvazione del federalismo municipale, che diventerà presto legge; oppure ricordiamo il lavoro della Commissione bicamerale sul federalismo regionale, che è altrettanto importante e che riguarda la vita di tutti noi: i soldi devono rimanere sul territorio e devono finire gli sprechi pubblici. Diamo finalmente al nostro Paese una speranza nuova, un fisco nuovo e una riforma fiscale, che tutti aspettano da anni. È su tali temi che chiamiamo l'opposizione al confronto. Lavoriamo insieme per cambiare questo Paese. Lo dobbiamo ai nostri precari, ai nostri figli, alle nostre famiglie, ai nostri giovani e ai nostri anziani; lo dobbiamo a chi ci ha dato il voto per riformare e cambiare questo Paese in meglio, in meglio, e non per farlo rimanere sempre fermo al palo. Lavoriamo per rendere questo Paese finalmente moderno. Signor Presidente, la Lega voterà a favore, per i contenuti e per i fatti positivi che il decreto-legge in esame

l'Italia e il Parlamento italiano devono ringraziare il Presidente della Repubblica italiana, perché sta nel suo impegno, nel suo rigore e nel suo equilibrio se ancora risuonano nel teatro istituzionale le parole e la forza della Costituzione e della legge, e se esse producono fatti. Ho sottolineato l'espressione «se producono fatti», perché gran parte delle osservazioni contenute nelle lettere inviate dal presidente Napolitano ai Presidenti di Camera e Senato erano state comunque oggetto di discussione in quest'Aula, di nostre pregiudiziali di nostri interventi. Ma, come sappiamo, questo non è luogo che abbia orecchie attente, appunto, ad obiezioni e a rilievi che nella Costituzione e nella legge affondino le loro ragioni. Certo, c'è da capirlo, visto che il presidente Berlusconi, proprio qualche giorno fa, esattamente il 23 febbraio, è tornato ad insistere pubblicamente sui troppi vincoli legislativi che frenano l'azione di governo, ma in particolare sul fatto che il suo Esecutivo è un focoso destriero purosangue purosangue che - *sic* - viene appesantito dal Parlamento e dal Quirinale, diventando così un lento e impacciato ippopotamo; e ancora, sulle prerogative del Quirinale, per esempio,

un atto di irresponsabilità, naturalmente, nel momento in cui peraltro ha accusato il Parlamento di rendere un ippopotamo il figlio di quel destriero purosangue che era il decreto originario, e anche di mistificazione, perché qualunque persona di buon senso che stia alla realtà dei fatti sa bene che il maxiemendamento censurato dal Presidente della Repubblica era stato partorito dal ventre di quel destriero purosangue, ed era suo figlio legittimo. È questa la ragione per la quale, signor Presidente, noi riteniamo di annunciare qui che il Gruppo del Partito Democratico presenterà un disegno di legge che renda costituzionale la norma dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 che impone che il contenuto dei decreti-legge sia omogeneo e corrispondente al titolo. una norma che è stata più volte esaminata dalla Corte costituzionale e invocata da diversi Presidenti della Repubblica, alla quale vogliamo dare il vigore, la forza di una norma costituzionale, sperando così che non venga ancora una volta spazzata via dal campo di quelle che vengono ritenute inutili questioni sollevate dal Parlamento, se il presidente Berlusconi, dopo la sua approvazione, avrà ancora il timone del Governo del Governo di questo Paese. Voglio spiegare ai cittadini italiani che facciamo questa operazione perché solo un potere che sta dentro le regole, che si muove secondo le regole e che obbedisce alla legge è un potere che può essere controllato dai cittadini e che i cittadini possono, dunque, verificare nel suo operato. Ora abbiamo di fronte questo decreto-legge che, sia pure amputato in qualche parte, è comunque il frutto deforme - senza padre e senza madre, perché tutti, improvvisamente, ne disconoscono paternità e maternità - di di questa legislatura e di questo Governo. Io ripercorro molto brevemente le misure contenute in questo decreto-legge, perché interesseranno i cittadini italiani che ci ascoltano, ed è giusto che essi sappiano. Con questo decreto aumentano le tasse: aumenta la tassa sui rifiuti, la tassa sull'energia e sulla benzina; si introduce la tassa sul cinema. Si crea la tassa della disgrazia, per cui i cittadini che abitano in un territorio che subisce una calamità naturale, anche gravissima, pagheranno loro stessi i danni di quella calamità naturale. Eppure questo Paese, che aggiunge tasse, come diceva oggi il Governatore della Banca d'Italia,

Le banche vincono la battaglia sulle somme illegittimamente addebitate sui conti correnti e si aggira il conflitto di interesse. Io qui voglio dire che quanto detto poc'anzi dal presidente Gasparri non è esatto anzi, è profondamente sbagliato. Infatti, la stesura approvata in prima lettura dal Senato non era una proroga del divieto, ma era una ipotesi ordinamentale, piuttosto pasticciata, che aveva l'obiettivo principale di bloccare le ipotesi espansive del concorrente di Mediaset, Quell'ipotesi era fondata, peraltro, anche su un aumento di un'altra invenzione del presidente Gasparri, il cosiddetto SIC, il sistema integrato delle comunicazioni, che con il decreto milleproroghe francamente non c'entrava assolutamente nulla.

a vari capitoli si spesa, tra i quali la benzina per le auto dei Carabinieri e della Polizia di Stato. Insomma, alla fine, ci si è accontentati di cinque milioni di euro per quegli allevatori truffatori!

milioni per i truffatori tolti ai malati di cancro! Allora, quella invocazione «Roma ladrona», che risuona continuamente nei comizi della Lega Nord - lo dico ai cittadini italiani che ci ascoltano e a quest'Aula -francamente risulta assai beffarda e, soprattutto, falsa e menzognera.

in questo Paese quella che io, ormai, vedo schiettamente: una separazione sempre più evidente tra l'Italia com'è, cioè l'Italia bella, l'Italia bella, e una maggioranza e un Governo che, un po' con la «legge porcata» e i suoi effetti, e un po' con le capacità seduttive (chiamiamole così) del presidente Berlusconi, tengono il potere. Certo è frenetico: infilano nel primo provvedimento che passa tutto quello che possono, fino all'ultimo morso, per mordere, fino a quando possono, un poco di polpa dall'osso che gli è stato consegnato con il governo del Paese. Ma io credo che questo tempo stia passando, che l'Italia

solidarietà - e credo di trovare la condivisione dell'intera Aula - nei confronti della battaglia del popolo libico, che in questo momento è oggetto di un'operazione di grande sterminio.

La democrazia è un bene prezioso, la democrazia è un bene inviolabile, la libertà dei cittadini è un bene sacro e non potrà mai essere censurata o impedita con azioni di forza, con azioni violente, con azioni cruente quali quelle a cui stiamo assistendo e alle quali credo, a breve, la comunità internazionale riuscirà a dare le opportune risposte. Mi auguro che, al più presto, sia l'Unione europea che la comunità internazionale sappiano individuare quelle scelte e quelle strategie per evitare che tale sterminio continui. La democrazia è sacra, e siamo anche noi chiamati ad invocarla e a difenderla, anche per i nostri amici del popolo libico.

i senatori del Popolo della Libertà esprimeranno il loro voto favorevole al provvedimento in esame. Prima di iniziare la dichiarazione di voto, voglio però ringraziare i relatori il presidente della Commissione bilancio Azzollini, con cui abbiamo lavorato, nonché tutti i componenti delle Commissioni, che di giorno, di pomeriggio e anche di notte hanno lavorato per portare in Aula, due volte, questo provvedimento. È stato un dibattito difficile da gestire. Abbiamo discusso di 1.550 emendamenti oltre alle riformulazioni degli emendamenti che erano stati dichiarati inammissibili e ai subemendamenti operando però un confronto ampio che ha visto maggioranza e opposizione incontrarsi spesso sugli emendamenti per dialogare e verificare possibili elementi su cui concordare, al di là del voto finale, che ovviamente si è diversificato, ma non si può dire così del lavoro che è stato compiuto insieme. Non farò l'elenco già lungamente riproposto, anche se vorrei ricordare, al di là delle cose estremamente negative che ho sentito in Aula, che con questa legge si finanziano il 5 per mille e le reti di energia, si dà risposta agli alluvionati di varie Regioni del nostro Paese, si danno fondi all'editoria,

alla proroga del divieto di incroci tra le televisioni e la stampa, è bene ricordare due In primo luogo, la legge Gasparri, che ha fissato questi principi, è l'unica legge in materia mai impugnata da nessuno di fronte alla Corte costituzionale, in un settore delicato che ha visto la Corte intervenire su quasi tutti i provvedimenti in questa materia.

Siete stati al Governo e non avete spostato il termine; siete andati all'opposizione, e pretendete che il termine venga spostato. È un po' come il conflitto di interessi: quando governate non ve ne occupate, quando siete all'opposizione ci dite che bisogna occuparsene. *(Applausi dai Gruppi Tutto questo avviene per un problema di difficoltà oggettiva nei rapporti tra le nostre istituzioni,

Questo è il tema che dobbiamo affrontare, senza primi della classe che qui, in questa Aula, non ci sono in alcun Gruppo politico. Voglio ricordare, a chi ha parlato del mostro che abbiamo generato in quest'Aula del Parlamento, che il Governo ha presentato

Il collega sa bene, essendo stato in Commissione, chi ha approvato i singoli articoli e chi ha approvato il provvedimento globale. Ma vorrei ricordare proprio al collega che mi ha interrotto che nel 2008, *in articulo mortis*, il Governo presieduto dal professor Prodi in Parlamento modificò il cosiddetto milleproroghe aggiungendo 56 articoli e 169 commi, di cui 70 non erano né proroghe né disposizioni urgenti in materia finanziaria. *(Applausi che il nostro provvedimento viene dopo una legge di stabilità fatta di 71 commi, mentre il provvedimento di quel Governo venne sette giorni dopo una finanziaria di 1.193 commi. E se non bastasse quel che ho detto per far capire di cosa stiamo parlando, vorrei ricordarvi che quel provvedimento, sotto legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria», si occupava di: modifiche del codice della proprietà industriale; inquadramento *ope legis* dei dirigenti penitenziari; norme sulla responsabilità degli amministratori di società partecipate; deroga all'ordinamento giudiziario; aumento dell'indennità degli ispettori ENAV; finanziamento degli interventi alla caserma «Rossani» nel quartiere Carrassi di riordino dei consorzi di bonifica. E, udite udite, aumento della durata in carica dei membri della CONSOB, del Garante dei dati personali, dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e gli appalti. *(Applausi dal Gruppo PdL)*. Questo era il provvedimento del 2008, esattamente tre anni fa.

dobbiamo prendere atto che siamo ad un punto in cui la frammentazione ha superato il velo pietoso della cosiddetta teoria dell'omogeneità teleologica, abbandonandosi allo *ius singulare*. È questo il tema che dobbiamo affrontare. Vogliamo darci nuovi Regolamenti? Vogliamo nuovi ruoli per le Camere? Vogliamo dare nuove possibilità al Governo, che è eletto dalla maggioranza dei cittadini, di portare avanti il proprio programma in tempi certi, senza bisogno di fare decretazione d'urgenza? Se vogliamo farlo, possiamo farlo, ne abbiamo anche parlato in quest'Aula, ma non nascondiamoci dietro un dito come se fossimo Alice e questo fosse il Paese delle meraviglie! Questi sono problemi che conosciamo da anni e nei quali si sono imbattuti tutti i Governi; e l'elenco delle cose che ho fatto poc'anzi, che sono contenute in questo decreto, scontano un interesse per il Paese. come non è vero quello che qualcuno ha detto qui e nell'altro ramo del Parlamento, che abbiamo tagliato i fondi alla legislazione in materia di assistenza ai malati oncologici, che vengono aumentati di 40 milioni in un articolo di questa legge, e 100 milioni vengono dati per la cura della SLA. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).* Questo è l'impegno di questo Governo! Salvo che non si voglia pensare che tutto debba avvenire attraverso la strumentalizzazione dei principi della Costituzione, oggi su un decreto, usando la Costituzione come una clava per combattere il proprio avversario, e nei giorni scorsi dopo che il Governo aveva avuto la fiducia. Le opposizioni che hanno fatto? Il Governo prende la fiducia e invocano lo scioglimento anticipato, dimenticando che peraltro lo scioglimento anticipato non può essere attuato contro un Governo che gode della fiducia in tutti e due i rami del Parlamento. Ma sono quelle stesse forze politiche, colleghi dell'opposizione, che quando ci permettemmo di dire che se fosse venuta meno la maggioranza che ha dato al Parlamento questa maggioranza di deputati e senatori bisognava tornare alle urne, hanno detto: no, qualunque maggioranza si trovi in Parlamento, possiamo continuare a governare. Quindi, secondo questa Costituzione *à la carte*, se si ha la maggioranza e si prende la fiducia in Parlamento si deve andare ad elezioni, se si perde la maggioranza che è stata data dagli italiani invece si può trovare un'altra maggioranza per governare! *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).* Non ci stiamo a questa interpretazione delle regole, e vi diciamo che siamo pronti ad andare avanti governando nell'interesse del Paese, attuando le riforme che possono consentire al Parlamento di non perdere la centralità e al Governo di assolvere il proprio compito con il patto assunto nei confronti degli elettori, nei modi e nei tempi che interessano l'economia, la vita delle famiglie e la vita delle imprese. Per queste ragioni, i senatori del Popolo della Libertà voteranno a favore di questo provvedimento e metteranno mano dalle prossime settimane alla riforma della nostra Costituzione per aggiornare il modo di essere del Parlamento, del Governo e della vita istituzionale di questo nostro Paese.